«Cara Presidente, mi onoro informarLa che la Camera dei deputati, in data 24 marzo 2018, nella sua prima seduta, mi ha eletto Presidente e che, nella seduta ha avuto luogo il mio insediamento. Con stima e cordialità. F.to: A nome mio personale e di tutta l’Assemblea rivolgo al presidente Fico i più cordiali auguri di buon lavoro. (Applausi). Comunico inoltre di aver ricevuto la seguente lettera: «Roma, 24 marzo 2018 Onorevole Presidente, La informo che in data odierna ho rassegnato al Capo dello Stato le mie dimissioni. Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere e ha invitato il Governo a restare in carica per il disbrigo degli affari correnti. F.to: Paolo Ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento, le senatrici e i senatori hanno indicato alla Presidenza i Gruppi parlamentari dei quali intendono far parte. In allegato al Resoconto della seduta odierna sarà pubblicato l’elenco dei componenti di ciascun Gruppo. In data 27 marzo i Gruppi parlamentari hanno proceduto alla loro costituzione. Gli Uffici di Presidenza risultano essere così composti: Gruppo MoVimento 5 Stelle Presidente: Toninelli Vice Presidente vicario: Crimi Vice Presidenti: Moronese, Patuanelli, Perilli, Pesco Segretari: Castaldi, Puglia, Santangelo Tesoriere: Catalfo Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente Presidente: Bernini Gruppo Lega-Salvini Premier Presidente: Centinaio Vice Presidente vicario: Candiani Vice Presidenti: Stefani, Solinas, Borgonzoni Tesoriere: Borghesi Gruppo Partito Democratico Presidente: Marcucci Gruppo Fratelli d’Italia Presidente: Bertacco Gruppo Misto Presidente: De Petris Vice Presidenti: Buccarella, Nencini Gruppo Per le Autonomie (SVP-PATT, UV) Presidente: Unterberger La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha stabilito all’unanimità che, ai sensi dell’articolo 24 del Regolamento, sia nominata una Commissione speciale per l’esame degli atti urgenti presentati dal Governo. In conformità ai precedenti, la Commissione speciale sarà composta da 27 membri in rappresentanza proporzionale su designazione dei Gruppi. Oltre ad avere la competenza di merito sui singoli provvedimenti, assorbirà le competenze di ogni altra Commissione in sede consultiva, anche con riguardo agli eventuali pareri obbligatori. I Gruppi parlamentari provvederanno a designare i propri rappresentanti nella Commissione speciale entro le ore 12 di domani, giovedì 29 marzo.

reca: «Votazione per l’elezione dei quattro Vice Presidenti, dei tre senatori Questori e degli otto senatori Segretari». Ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento, ciascun senatore scriverà sulle proprie schede, rispettivamente, due nomi per l’elezione dei quattro Vice Presidenti; due nomi per l’elezione dei tre senatori Questori; quattro nomi per l’elezione degli otto senatori Segretari. Saranno eletti coloro che otterranno il maggior numero di voti. Al fine di prevenire ogni possibile equivoco, è a disposizione dei senatori l’elenco dei colleghi che hanno lo stesso cognome, con l’indicazione dei rispettivi nomi. Per semplificare lo svolgimento delle operazioni di voto, sono state predisposte due cabine. I colleghi senatori transiteranno sotto il banco della Presidenza per depositare le proprie schede nelle tre distinte urne collocate all’uscita di ciascuna delle predette cabine. La chiama sarà svolta in ordine alfabetico. Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento, procedo al sorteggio degli otto componenti della Commissione di scrutinio, addetti allo spoglio delle schede.

Di Marzio, Magorno,

Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori componenti la Commissione di scrutinio a procedere allo spoglio delle schede, che avverrà nell’adiacente Sala Pannini. In attesa dei risultati della votazione, sospendo la seduta.

dei senatori Segretari. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto per l’elezione dei quattro Vice Presidenti:

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto per l’elezione dei tre senatori Questori: presenti 315 Senatori votanti 314 Hanno ottenuto voti i senatori: De Poli 165 Arrigoni 130

Pisani Giuseppe 104 Margiotta 63 Nastri 18 De Poli 2 Bressa 1 Di Micco 1 Lupo 1 Santanchè 1 Urraro

A nome dell’Assemblea e mio personale, desidero rivolgere ai Vice Presidenti, ai senatori Questori e ai senatori Segretari eletti il più cordiale augurio di buon lavoro. (Applausi).

Il Senato è convocato a domicilio. La seduta è tolta